In merito alla questione relativa alla chiusura del traffico aereo civile dell'aeroporto di Trapani Birgi e alle conseguenti problematiche per i settori produttivi locali, l'Amministrazione della Difesa - ed in particolare l'Aeronautica militare (AM) - ha dimostrato, fin da subito, grande sensibilità e soprattutto piena disponibilità nella ricerca e nella individuazione di una soluzione che fosse in grado di contemperare le prioritarie operazioni militari in corso connesse alla nota emergenza libica con le esigenze del traffico civile. Infatti, l'Aeronautica militare ha ricoperto un importante ruolo strategico, svolgendo un'incisiva e costante funzione di raccordo con tutte le parti in causa - ENAC, ENAV,

ha consentito, sia pure con le limitazioni correlate alle operazioni militari, già a partire dal 30 marzo scorso l'apertura parziale al traffico commerciale, con la messa a disposizione, per le esigenze dello scalo civile, di quattro piazzole di sosta, anche notturna, nonché di 36 *slot*

L'accordo tecnico, dunque, costituisce di per sé un risultato molto importante, se si pensa alla delicatezza e alla complessità della situazione ed anche alle molteplici e variegate difficoltà che è stato necessario superare prima di poter assicurare il ripristino parziale del traffico aereo civile. Occorre precisare che l'attuale indeterminatezza della situazione non consente di stabilire con certezza il momento per la riapertura totale dello scalo al traffico civile, che rimane comunque un obiettivo. Si assicura, tuttavia, che l'Aeronautica militare è intenzionata a proseguire, nel solco della disponibilità offerta fin dall'inizio di tale esigenza, a valutare il progressivo incremento del numero dei voli civili, compatibilmente con l'evolversi della situazione e le necessità della difesa aerea e quelle derivanti dagli impegni internazionali assunti dal nostro Paese. Devo sottolineare che il raggiungimento di criteri operativi indispensabili a mantenere la piena operatività sia dell'attività militare che di quella civile sull'aeroporto di Trapani deve tenere conto: dell'indispensabile capacità di assicurare il livello di sostegno logistico adeguato alle complesse operazioni in corso; del mantenimento delle misure di sicurezza per la componente necessarie per la presenza sull'aeroporto di intenso traffico militare al massimo livello di operatività; delle esigenze di ridurre i rischi di congestione dei voli commerciali in arrivo e partenza per poter assicurare la giusta separazione dei traffici sulle piazzole e in volo in coerenza con le regole del traffico aereo. se può apparire superfluo, desidero, comunque, sottolineare le ragioni alla base della decisione iniziale di chiudere lo scalo

Sottolineo in proposito che l'aeroporto di Trapani-Birgi, come è noto, ai sensi del decreto ministeriale del 25 gennaio 2008, è un aeroporto militare destinato al ruolo di *Deployment Operating Base* Ciò significa che l'eventuale apertura al traffico aereo civile é subordinata al rispetto di determinate condizioni, in particolare quella secondo cui «l'operatività della base e le esigenze militari rivestono aspetto prioritario su ogni altra attività e, pertanto, limitazioni potranno essere comunicate anche con brevissimo tempo di preavviso». la decisione della chiusura dell'aeroporto al traffico aereo civile, presa il 20 marzo scorso, con il massimo di preavviso oggettivamente possibile ed in stretto coordinamento con ENAC ed ENAV, è riconducibile alla necessità di garantire lo svolgimento di tutto il complesso di attività militari connesse all'operazione in atto, evitando tutti i possibili rischi,

Un ulteriore elemento che contribuisce ad indicare la misura dell'intensità dell'attività complessivamente effettuata presso tale aeroporto va rilevata nel fatto che su tale base, oltre al traffico militare - nazionale ed

Infine, con riferimento al quesito relativo alla scelta delle basi militari per il supporto delle operazioni aeree in corso, faccio osservare che la scelta per l'uso della base di Trapani determinata da una perfetta combinazione dei fattori più influenti ai fini delle predette operazioni, che sono costituiti evidentemente dalla sua dislocazione geografica molto prossima all'area di interesse, nonché dalle capacità logistiche, in termini di aree di parcheggio, stoccaggio dei materiali ed armamenti, rifornimenti,

sugli aspetti relativi al settore turistico-alberghiero, che ha subito l'impatto delle operazioni in corso. Tenuto conto che la fruizione di sistemi di trasporto efficienti e prossimi alle zone in cui sono presenti strutture ricettive turistiche è una evidente esigenza prioritaria per il mantenimento dei flussi di presenze e per lo sviluppo del settore, si conferma l'auspicio che la situazione possa evolvere a breve in modo da attuare il ripristino graduale dell'attività commerciale sul sedime di Trapani Birgi, evitando ulteriori pesanti penalizzazioni per turisti ed operatori. Il Governo guarda, con la massima attenzione e sensibilità, al tessuto imprenditoriale trapanese, nella consapevolezza che l'industria turistica rappresenta per l'economia della Sicilia, e per la provincia in questione in particolare, un *asset* fondamentale, quale settore propulsivo del sistema economico di un'isola che fa delle sue bellezze naturalistiche ed artistico-culturali un punto di forza distintivo e che va quindi difesa anche mediante l'individuazione di efficaci sinergie con la Regione siciliana, cui sono riservate, anche in virtù dello Statuto speciale, incisive prerogative di intervento. Il Governo già si Il Governo già si era fatto carico di formulare un ampio programma di interventi a favore del turismo nel Mezzogiorno, con specifico riferimento al territorio dell'intera Sicilia in particolare. il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, quale organismo intermedio delegato nell'ambito del Programma operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo», cofinanziato dai fondi strutturali della Unione europea nella presente programmazione 2007-2013, sta elaborando un articolato programma promozionale relativo ai territori interessati da detto programma, tra cui diverse aree della Sicilia. L'azione di promozione, in linea con la strategia del programma, punta a valorizzare proprio l'offerta turistico-culturale e turistico-ambientale del Mezzogiorno ed utilizza varie tipologie di intervento e diversi strumenti operativi. L'azione promozionale è altresì accompagnata da iniziative di promo-commercializzazione delle offerte turistiche dei territori, alla luce anche delle positive ricadute economiche e occupazionali che lo sviluppo del turismo garantisce. Per il potenziamento dell'offerta turistica sono stati altresì destinati otto milioni di euro per interventi volti a rafforzare ed implementare il turismo regionale con gli obiettivi di realizzare itinerari enogastronomici e di qualificare l'offerta turistica legata al gioco del golf. Ai finanziamenti possono accedere gruppi di Regioni attraverso la presentazione di un progetto da realizzare. Inoltre, si segnala che sono previsti circa 112 milioni di euro per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale. Le risorse, che sono destinate a tutte le Regioni italiane, comprese quelle del Mezzogiorno, sono finalizzate alla realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale ed il recupero della sua competitività sul piano internazionale. Il Governo, pertanto, è nella piena consapevolezza della grave situazione venutasi a creare a Trapani, che ha ingenerato legittime preoccupazioni in ordine ai potenziali riflessi economici ed occupazionali correlati alla chiusura dello scalo A questo scopo, esso sta analizzando nell'immediato le modalità per l'inserimento, già nel prossimo provvedimento legislativo d'urgenza che riguarderà le missioni internazionali (con particolare riguardo alle operazioni in Libia), di disposizioni che prevedano interventi di ristoro per le popolazioni e misure compensative di sostegno e di rilancio da attuare a favore dei settori economici interessati, attualmente valutabili nell'ordine di 10 milioni di euro. Il Dicastero della difesa, in particolare, proseguirà a seguire con la massima attenzione l'evolversi della situazione, nella prospettiva di riaprire con gradualità lo scalo di Trapani in maniera totale, non appena le condizioni lo renderanno possibile.

parzialmente soddisfatto. Infatti, la sollecitazione che è venuta da tutti i parlamentari siciliani, di maggioranza e opposizione, rispetto ad una scelta assunta in condizioni di necessità, cioè l'utilizzo immediato

Pertanto, l'idea che oggi una parte degli usi civili dell'aeroporto sia stata ripristinata è qualcosa che valutiamo positivamente e ne prendiamo atto con soddisfazione.

innanzitutto, non riguarda solo la liquidazione in forma compensativa di un danno di immagine che Trapani e la Sicilia hanno riportato, e che continuano a riportare, dalla vicenda dell'aeroporto di Trapani a tutte le vicende che hanno riguardato e continuano a riguardare Lampedusa, Mineo e così via. Consideriamo, infatti, che vi è una serie di risorse, quali, ad esempio, i fondi FAS, che sono nella disponibilità del Governo ma che sono bloccate, mentre potrebbero essere destinate, ad esempio, nella rimodulazione del POR 2007-2013, al completamento della seconda pista di atterraggio proprio dell'aeroporto civile di Trapani, condizione che rappresenterebbe un volano di sviluppo molto più ampio e più consistente di una campagna promozionale

non ci è stato detto perché - e dal punto di vista tecnico-militare non credo sia un segreto - la base di Comiso o quella di Sigonella non possono essere utilizzate di più per gli scopi militari permanenti che comportano le scelte del nostro Governo e la nostra

Però, signor Sottosegretario, bisogna specificare un ulteriore elemento. È vero che lo scalo aereo di Birgi è nato come scalo militare, ma in particolare negli ultimi anni, grazie ad investimenti di milioni di euro, è diventato soprattutto uno scalo civile.

ritengo soddisfatta se parzialmente adesso si riesce a coprire quasi il 70 per cento dei voli; però dobbiamo considerare che nel mese di agosto, grazie al e all'offerta che l'aeroporto ha dato a tutta l'Europa, avremmo coperto con i voli circa 88 movimenti giornalieri, cioè 44 voli al giorno.

quando è stata immaginata la nuova stagione primaverile ed estiva. Speriamo che si possa presto avere la riapertura totale del traffico.

deviazione dell'indirizzo degli sbarchi di extracomunitari rispetto alla destinazione prevalente di Lampedusa. Abbiamo quindi da ristorare, non soltanto, e principalmente, i lavoratori, 150 dei quali oggi hanno

L'aeroporto di Trapani Marsala Birgi in quattro anni ha quintuplicato le sue presenze: dai 300.000 passeggeri del 2006

quindi tutti utili ad alimentare un obiettivo di sviluppo turistico del territorio che ha fatto della Provincia di Trapani l'unica che negli ultimi quattro anni ha segnato un incremento delle

per essersi seduti immediatamente attorno ad un tavolo per verificare, al di là di quelle che potevano apparire condizione proibitive, le possibilità di riattivare lo scalo civile. Per questo voglio ringraziare personalmente anche il sottosegretario Cossiga, che ha subito individuato la gravità delle conseguenze che potevano derivare in capo al territorio trapanese dal perdurare della chiusura dell'aeroporto. ma sempre con la massima attenzione, come del resto tutto il territorio trapanese ha fatto, mobilitandosi in una civile e silenziosa, ma determinata richiesta di immediata riapertura del suo scalo,

della Maddalena, ci tengo assolutamente a precisare che le stesse sono totalmente prive di fondamento, come peraltro dichiarato con nota ufficiale del 5 aprile scorso dal Comando militare marittimo autonomo della Sardegna, organo istituzionalmente responsabile della gestione e dell'operatività della Marina militare in tutta l'isola. Si è trattato di un crescendo di informazioni che, partite forse come una specie di pesce d'aprile, poi sono state corredate da una serie di

Non posso che confermare quanto riportato dall'Ente militare, ossia che nell'arcipelago non c'è stato alcun sopralluogo, né di ufficiali americani né di personale dell'Amministrazione della Difesa statunitense, che non è mai stato ipotizzato un ritorno delle navi americane a Santo Stefano

del Governo, perché non nascondo - non ve ne sarebbero motivi - di aver salutato tre anni fa la partenza degli americani con un sentimento di sollievo, di soddisfazione e, per certi versi, anche di gioia. La perentorietà della risposta fornita dal sottosegretario Cossiga mi pare non lasci adito a dubbio alcuno.

vorrei consegnare alla sua attenzione la preoccupazione che si diffonde in Sardegna, in generale, e nell'ambito gallurese, in particolare

che quella comunità attende in relazione all'utilizzo trentennale che del territorio è stato fatto per fini militari. Si era parlato di riconversione. Era stata anche individuata La Maddalena come località nella quale svolgere e celebrare il G8. Poi si è ritenuto di dover andare altrove, ma soprattutto, e questo costituisce motivo di preoccupazione, oltre che di sofferenza per quella comunità, di dover utilizzare la Maddalena come palestra nella quale esercitare soprusi e angherie compiuti in nome della realizzazione di un grande evento ad opera della Protezione civile, carpendo la buona fede di quelle popolazioni e sottraendo le risorse che avrebbero dovuto dovuto essere impiegate altrimenti. Consapevole della sensibilità del Sottosegretario, lo esorto affinché possa esperire tutti i tentativi nei confronti del Ministro della difesa, della cui sensibilità in verità non ho altrettanta sicurezza, e, soprattutto, nei confronti dell'intero Gabinetto,

Vorrei infine, ringraziando la Presidenza anche per questa ulteriore cortesia, sottolineare che il timore che potesse esserci un ritorno alla militarizzazione è figlio di una situazione sarda particolarmente delicata. Il 60 per cento delle servitù militari italiane è sistemato nella Regione Sardegna in questa stagione, piuttosto che assistere ad un ritorno di quanti erano già andati via, vorremmo non solo vedere confermata, come stasera è accaduto, la partenza degli americani, ma magari anche, in un quadro di risanamento e di bonifica del territorio, recuperare altre aree, delle quali il Senato, alla presenza dello stesso

di chiedere al Sottosegretario ciò che non gli verrà certamente difficile, cioè di continuare a lavorare affinché questo 60 per cento si riduca gradualmente, perché, come si dice in tutte le parti d'Italia, «noi abbiamo già dato».

Grazie della quale era previsto tutto uno scadenzario di impegni da parte del fondo svizzero GITA, che doveva subentrare nell'operazione. Nessuna delle scadenze è stata rispettata. Oggi sono a rischio 450 posti di lavoro. I lavoratori sono molto preoccupati, ma c'è una preoccupazione che va al di là dei posti di lavoro che si perdono (che non sono nemmeno una cifra esorbitante, anche se dietro ognuno di quei posti c'è comunque una famiglia, una professionalità ed un lavoro svolto per anni al servizio Grazie Il Governo in questi mesi ha seguito la questione e ha preso anche degli impegni. Leggo testualmente la dichiarazione rilasciata dal ministro Romani a Porto Marghera,

che si produce appunto negli stabilimenti che ho prima citato, è la terza produzione di materia plastica nel mercato mondiale: quindi, è una produzione strategica per l'industria chimica e per l'intero ciclo manifatturiero. La materia prima della filiera del PVC proviene dal *cracking*, che in Italia è presente nei petrolchimici di Marghera, Priolo, Brindisi e, appunto, Porto Torres. Se sparisse la filiera del cloro-PVC, detenuto in Italia principalmente dalla Vinyls, si creerebbe un disequilibrio in tutti i distretti chimici del Paese.

l'Italia in qualche modo è uscita dalla chimica, perché all'inizio degli anni '90, con un processo di ristrutturazione molto profondo, che ha toccato in particolare Enichem, ma non soltanto, è rimasta molto marginale rispetto alla produzione della chimica,

Dopo due anni di tira e molla, sembrava che negli ultimi giorni, alla fine di marzo, si fosse trovata la via d'uscita, e il fondo GITA si era impegnato a fare il versamento dei 100 milioni che servono per fare l'operazione, i 100 milioni a tutt'oggi non sono stati versati. Cominciano ad essere a rischio gli stipendi, e voglio ricordare che le forme di lotta hanno raggiunto livelli esasperati, i lavoratori sono stati per lunghi periodi sulle ciminiere, c'è una situazione molto preoccupante.

ogni vertenza viene seguita come se fosse una vertenza a parte, non la si affronta in un contesto complessivo come dovrebbe essere quello della chimica. Continuando in questo modo si perdono dei pezzi di produzione e via via si impoveriscono il sistema produttivo e l'industria italiana. italiana. Vi chiedo uno sforzo, perché non si salva soltanto il posto di quei 450 lavoratori e di tutto l'indotto, ma si salva un importante pezzo di industria del nostro Paese, che negli anni '90 era un'industria d'avanguardia,

della Cassa depositi e prestiti e della possibilità che essa svolga un ruolo di intervento anche nella ripresa dell'industria nel nostro Paese. Credo che anche da questo punto di vista andrebbe una riflessione appunto per affrontare il problema della reindustrializzazione del Paese. Credo quindi che sia giunto il momento di dire, su questa vertenza, una parola chiara per i tanti lavoratori e per il futuro di questo settore.

Signora Presidente, ritengo utile ricostruire, ai fini di un'esauriente risposta ai senatori interroganti, la vicenda di Vinyls conseguente alla dichiarazione di insolvenza che ha portato al commissariamento della società. È noto infatti che la crisi di questa impresa chimica, che produce prevalentemente PVC, ha origine dalla decisione della multinazionale inglese INEOS, già nel 2007, di dismettere i propri impianti di produzione. Fatta questa precisazione, si ritiene utile ricostruire puntualmente quanto avvenuto, a partire dal fallimento della società e dalla successiva decisione del tribunale di Venezia, avvenuta in data 7 agosto 2009, di dichiarare l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla Vinyls spa. Il 13 agosto 2009 sono stati nominati dal Ministro dello sviluppo economico i commissari straordinari della citata società, già commissari giudiziali. In data 20 novembre 2009, i commissari straordinari della Vinyls hanno depositato il programma della procedura, che prevede la cessione dei complessi aziendali. Il 20 gennaio 2010 essi hanno depositato il documento integrativo al programma di cessione nel quale viene quantificato il fabbisogno finanziario necessario per il riavvio degli impianti, stimato in circa 30 milioni dì euro, per il quale i commissari intendono chiedere la garanzia del Tesoro. Con decisione del 25 marzo 2010, la commissione UE ha concluso l'istruttoria precisando che la concessione del prestito garantito dal Tesoro a favore di Vinyls Italia spa è compatibile con il mercato unico. Nel frattempo, a seguito della pubblicazione sui quotidiani di un invito a manifestare interesse all'acquisto della società menzionata, è pervenuta una sola risposta, da parte della RAMCO, gruppo del Qatar. La trattativa con il gruppo del Qatar tuttavia non è andata a buon fine e, di conseguenza, la RAMCO ha ritirato la propria proposta. Con decreto in data 8 giugno 2010 è stata approvata l'esecuzione del programma di cessione presentato dai commissari. Il 22 luglio 2010 è stato siglato il protocollo d'intesa ENI-Ministero dello sviluppo economico, in base al quale l'ENI si è resa disponibile a cedere gli *asset* necessari per garantire agli eventuali interessati la realizzazione dell'integrazione del ciclo del cloro. Anche sulla base della disponibilità acquisita da ENI a favorire la ricomposizione del ciclo del cloro, nel mese di settembre 2010 e stato pubblicato un bando di gara internazionale per l'acquisizione di offerte di acquisto. All'esito della pubblicazione del bando di gara, sono pervenute presso il notaio incaricato le seguenti offerte: offerta GITA Holding AZ, fondo svizzero, avente ad oggetto tutti e tre gli stabilimenti, condizionata all'acquisizione degli *asset* ENI, ai fini dell'integrazione del ciclo del cloro (in particolare, l'offerente GITA propone di acquistare i complessi aziendali tramite una *newco*,

avente ad oggetto i siti di Ravenna e Porto Torres; offerta IGS-industrie generali spa, avente ad oggetto il solo impianto PVC di Ravenna. Con relazione del 9 novembre 2010, i commissari straordinari, nell'esprimere un giudizio di preferenza per l'offerta GITA, hanno manifestato la necessità di rinviare ogni definitiva valutazione alla verifica della possibilità che venga rimossa la condizione apposta all'offerta medesima, e cioè l'acquisizione degli *asset* ENI. Nelle more della conclusione delle trattative tra GITA ed ENI, il fondo svizzero, al fine di consentire a Vinyls di far fronte alla difficile situazione finanziaria, si è impegnato all'acquisto di materia prima giacente presso gli stabilimenti Vinyls. Questo impegno, ad oggi, non è stato onorato. Il 1° marzo 2011 è stato siglato il contratto tra ENI, attraverso la Sindyal e Vinyls Group (la *newco* costituita da GITA per gestire l'operazione), per la cessione degli *asset* di ENI, la cui efficacia è stata, però, subordinata alla preannunciata capitalizzazione della *newco* per 100 milioni di euro. In conseguenza di questo vincolo, i commissari hanno invitato GITA a procedere alla capitalizzazione della *newco* per 100 milioni di euro, nonché a provvedere al pagamento del credito vantato, di cui ho detto, per l'acquisto della giacenza per circa 700.000 euro. Il Ministero dello sviluppo economico sta sostenendo, fin dall'inizio e nei limiti fissati dalla legge l'operato dei commissari, e segue con grande attenzione l'evoluzione della vicenda. In particolare, sta sollecitando, con un'adeguata azione di *moral suasion*, la conclusione delle procedure finanziarie che dovrebbero portare alla capitalizzazione di Vinyls Group. A questo proposito, non si può negare che qualche elemento di perplessità sta suscitando il comportamento del fondo GITA. I suoi continui rinvii, accompagnati da annunzi formali ai quali non seguono comportamenti concreti, non aiutano certamente a creare quel clima di collaborazione che è necessario al rilancio di un'importante impresa chimica. Si tenga presente, in proposito, che il piano industriale alla base dell'offerta di GITA prevede importanti investimenti che interessano tutti i siti, ma soprattutto quello di Porto Marghera. È quindi evidente qualora nei prossimi giorni - come comunicato dai commissari ai diretti interessati - non si verificassero i finanziamenti annunziati, si dovrà procedere all'esame delle altre offerte pervenute. Infine si ritiene utile precisare che il Ministero del lavoro, per quanto di propria competenza, ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti Vinyls per il periodo dal 23 novembre 2010 al 7 giugno 2011. Il trattamento è stato autorizzato per un numero massimo di 176 lavoratori della sede di Venezia, 101 lavoratori della sede di Porto Torres e per 35 lavoratori della sede di Ravenna.

(non si sa bene infatti per quali ragioni questi fondi avanzino delle offerte, visto che dietro non hanno un sistema produttivo e delle imprese),

Dispiace che nel corso di questa vicenda siano state fatte molte dichiarazioni da parte del Ministro, che in più di un'occasione ha suscitato l'illusione che la vicenda fosse vicina ad una conclusione.

soli. Tramite lei, sottosegretario Pizza, rivolgo un invito al Ministro affinché riprenda velocemente in mano la questione, la ponga all'interno del tavolo della chimica, convochi i sindacati, invii un messaggio preciso e puntuale ai lavoratori e cominci a valutare le altre offerte. Infatti, non ci si può far prendere in giro per

Se lasciamo andare avanti ancora questa questione, quegli impianti rischiano di depauperarsi in maniera irreversibile. Le forze lavoro migliori se ne andranno, dopo di che avremo fatto la frittata, senza dirlo e senza volerlo. Vi prego di prendere seriamente a cuore tale vicenda.

il 14 maggio 2010 la FILCAMS CGIL e la UILTUCS UIL, venute a conoscenza della pubblicazione della richiesta di partecipazione alla futura gara d'appalto per i servizi aggiuntivi presso i musei del polo fiorentino, hanno chiesto alla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della Città di Firenze di conoscere se era intenzione di quell'ufficio inserire una clausola di salvaguardia occupazionale per il personale dipendente dell'attuale concessionario Opera laboratori fiorentini. Il soprintendente ha provveduto immediatamente ad interessare della questione il responsabile unico del procedimento incaricato dell'istruttoria della gara d'appalto, informando contestualmente la direzione generale per la valorizzazione del Ministero, depositaria della stesura delle linee guida per la formulazione della gara e l'ufficio legislativo.

circa il fatto che le clausole di salvaguardia richieste sarebbero state inserite efficacemente nel bando vero e proprio nella misura consentita dalla normativa vigente, previo nulla osta della direzione generale per la valorizzazione, da predisporre nella seconda fase della gara ovvero dopo la scadenza delle richieste di partecipazione fissata il 15 settembre 2010. Dopo gli incontri fra il responsabile unico del procedimento e le organizzazioni sindacali del 9 settembre 2010, la Soprintendenza si è fatta latrice delle proposte della rappresentanza del personale di Opera laboratori fiorentini presso la direzione generale per la valorizzazione. È stato tuttavia rilevato che, nella tipologia di contratto nazionale di lavoro della Confcommercio il terziario la categoria della quale fanno parte i dipendenti del concessionario), non esiste l'obbligo per la stazione appaltante di inserire una qualsivoglia clausola di salvaguardia per i lavoratori. È stato quindi lo stesso Ministero a contattare la Confcommercio per sanare la situazione. Il 20 ottobre, tuttavia, le organizzazioni sindacali FILCAMS e UILTUCS hanno proclamato lo stato di agitazione che è sfociato, pur con le trattative in corso d'opera, nello sciopero degli addetti del 5 dicembre 2010. In data 10 dicembre 2010, presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali, è stato steso un protocollo d'intesa con Confcommercio settore terziario e le organizzazioni sindacali di categoria, cui ambito è stata redatta una clausola di salvaguardia occupazionale estesa anche ai contratti di lavoro del commercio che riguardano i concessionari dei servizi nei musei dello Stato. La Soprintendenza si è assunta l'impegno di inserire detta clausola nella documentazione relativa ai bandi di gara per servizi di ristoro, servizi di editoria e oggettistica e servizi integrati da essa banditi.

è stato fatto tutto ciò che era possibile fare - come lei giustamente ha detto - per risolvere il punto. Il problema però non è risolto. Ad oggi abbiamo 350 persone che non sanno cosa capiterà loro, perché i bandi non sono stati fatti, permane ancora una fase di incertezza

che verrà settorializzato l'intervento - che come lei sa è plurimo, in un'organizzazione come quella dei musei - finalizzato a singoli spezzoni di attività.

sancita, nel senso che l'unicità che oggi garantisce a musei importantissimi nel mondo di poter svolgere al meglio la loro attività verrebbe fatta saltare.

il Ministero per i beni culturali dia una risposta al quesito che i senatori hanno posto, perché in quello che lei ha detto questa risposta non c'è. Grazie lo stesso.

(ex lavoratori socialmente utili), si inserisce pienamente nei termini attuativi della direttiva ministeriale n. 103 del 30 dicembre 2010, concernente i contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie riconducibili alle funzioni previste per il profilo del collaboratore scolastico. riguardo, si riferisce quanto segue. Si premette che le spese per l'acquisto di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie nelle scuole rientrano nell'ambito, più generale, delle spese per il funzionamento delle medesime; rientrano, quindi, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche che, come è noto, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, fu istituito dall'articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, unitamente al Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato. Quanto alla suddetta direttiva n. 103 del 2010, con tale atto si è inteso fornire indirizzi per coordinare lo svolgimento dell'attività negoziale da parte delle singole scuole per l'acquisto dei servizi di pulizia loro eventualmente necessari. In attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, delle direttive comunitarie recepite col medesimo ed in accordo con la normativa sopra richiamata, la direttiva ministeriale citata non opera, né potrebbe, distinzioni tra le ditte che potranno partecipare alle procedure di acquisizione. In particolare, non si limita e non si potrebbe limitare la partecipazione alle sole ditte impieganti soggetti già titolari di progetti di lavoro socialmente utile od alle sole ditte già vincitrici di gare di appalto bandite dagli enti locali sino al 1998. Quanto sopra non pregiudica il fatto che si continuerà ad erogare le risorse finanziarie alle scuole per onorare tutti i contratti in essere, sino alla loro scadenza ed in attesa della conclusione delle procedure di gara (a cura delle scuole) per i nuovi contratti. I contratti in corso saranno onorati, ovviamente, indipendentemente dalla tipologia del personale dipendente dalle imprese svolgenti il servizio, comprese, quindi, le imprese che hanno stabilizzato (cioè assunto a tempo indeterminato) a suo tempo i soggetti già titolari di progetti di lavoro socialmente utile (cosiddetti ex lavoratori socialmente utili) o le imprese già titolari di contratti con gli enti locali o con le cooperative sociali di tipo B o, ancora, altre fattispecie comunque presenti. Va, inoltre, precisato che, nella direttiva del Ministro inviata alla Corte dei conti ed ancora in fase di registrazione, non sono definite le modalità di acquisto dei servizi che saranno effettuate secondo quanto previsto dal codice degli appalti. A tal fine l'amministrazione e la Consip hanno costituito un gruppo di lavoro, il cui compito è quello di predisporre uno strumento di acquisizione dei servizi di pulizia da rendere disponibile alle scuole nel più breve tempo possibile, indicativamente per l'anno scolastico 2012-2013. Nelle more della predisposizione di detto strumento, in assenza di convenzioni utilizzabili, le scuole, per acquistare i servizi, dovranno per forza avvalersi delle altre procedure, diverse dalla convenzione, rese disponibili dal codice dei contratti pubblici. La direttiva n. 103 del 2010 lascia alle scuole la scelta della procedura da utilizzare, in funzione delle specifiche necessità. Nel frattempo, il Ministero, per quanto attiene alle ripercussioni occupazionali, si è riservato di coinvolgere altri Dicasteri in modo da presentare una proposta congiunta alle organizzazioni sindacali dei lavoratori coinvolti. Per quanto attiene, infine, alla mancata retribuzione dei lavoratori, il Ministero ha assegnato alle scuole 260 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2010, somma già assegnata alle scuole per remunerare il servizio prestato dalle ditte in questione. Con tali somme nel corso dell'anno finanziario 2010 le scuole hanno saldato le fatture delle ditte sino al 31 del mese di agosto. Appena si sono rese disponibili le somme necessarie, il Ministero ha poi inviato alle stesse, vista la appostazione delle necessarie somme in bilancio, le relative risorse finanziarie per poter procedere al saldo delle rimanenti note contabili.

Nel frattempo, non abbiamo provveduto all'immissione in ruolo, e adesso i presidi si trovano in una stranissima situazione. Parliamo, infatti, di 14.000 persone che lavorano ormai da dieci anni nel mondo della scuola senza una contrattualizzazione definitiva e, tra le altre cose, con contratti a termine che risultano prorogati fino al 30 giugno. Capisco il sottosegretario Pizza, che ha fornito una serie di motivazioni, ma voglio ricordare allo stesso Sottosegretario che lo scorso gennaio

sospensione dei mesi di luglio e di agosto, senza copertura finanziaria. Non solo, ma è confermata anche l'applicazione della direttiva n. 103 del 30 dicembre 2010, che comporterà un taglio secco degli orari di lavoro, con una differenza di entità a seconda dell'esubero rispetto ai posti accantonati, con il 25 per cento di riduzione oraria in ciascuna scuola, e in alcune situazioni territoriali anche con tagli di posti di lavoro. Dalla stessa riunione, emerge anche il progetto del MIUR (che il Partito Democratico ha spesso contestato) secondo cui si vuole portare avanti un processo di esternalizzazione, con notevoli tagli di personale e salari, dovuti alla riduzione di finanziamenti, non più calcolati sul numero effettivo dei lavoratori ex LSU, ma sulla spesa equivalente agli abbattimenti del 25 per cento degli organici. Ciò ha significato, quindi che i presidi hanno dovuto prorogare i contratti scaduti al 30 giugno 2011 e mettere poi in fermo i lavoratori per luglio e agosto (a casa senza stipendio), tra l'altro senza alcun ammortizzatore sociale, e prevedere per l'anno 2011-2012 appalti provvisori in regime di cottimo fiduciario, cioè a trattativa privata: nella stessa trattativa privata, con decurtazione dei fondi, e peraltro senza tutelare il personale utilizzato. Ecco perché abbiamo presentato questa interrogazione. Aggiungo che non mi ritengo soddisfatta, perché significa tagli di posti di lavoro

Queste sono le domande che noi abbiamo posto, che tutti i presidi pongono, perché significa, da un lato, non tutelare i lavoratori che per 10 anni hanno garantito continuità di lavoro nelle nostre scuole, dall'altro non assicurare nè la pulizia nè la vigilanza delle aule scolastiche, e quindi, di conseguenza, non garantire alla scuola pubblica quei servizi che uno Stato, e soprattutto la nostra Costituzione, dovrebbero garantire. Per questo motivo non mi ritengo soddisfatta.

verrà data dal Senato particolare evidenza, anche con la pubblicazione sul proprio sito Internet, grazie ad una decisione assunta l'anno scorso, non risultano notizie non risultano notizie sulle dichiarazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale delle cariche direttive di alcuni enti specificamente menzionati nella legge n. 441 del 1982. Forse questo è dovuto ad una mia, oltre che degli organi di informazione, ma sarebbe interessante sapere chi ha presentato queste dichiarazioni e dove si possono trovare, perché, secondo la legge, andrebbero pubblicate in un apposito bollettino, di cui non si ha notizia.

finestra") del lontano 9 luglio 2009, riguardante le direttive che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve dare di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri per stabilire i criteri per la definizione di aree destinate al parcheggio

l'erogazione di multe nei confronti di coloro che non rispettano le norme fissate dai Comuni, sarebbe importante sapere quali sono queste direttive, perché anche queste non risultano reperibili, almeno dalle ricerche che io ho compiuto.